Onorevoli colleghi, due anni or sono, il 7 novembre, si spegneva a Milano, dopo una lunga malattia, la senatrice Alma Cappiello. Avvocato civilista, la sua autentica passione per la promozione e la tutela dei diritti di libertà delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, l'aveva spinta ad impegnarsi nella politica. Nel 1984 diviene coordinatrice della prima Commissione nazionale per le pari opportunità, istituita dal Governo Craxi, e l'anno successivo è eletta alla Camera dei deputati nelle liste del Partito Socialista; nel 1992 entra infine a far parte della nostra Assemblea. Il suo impegno parlamentare, vissuto con la tenacia e la concretezza che l'hanno sempre contraddistinta, fu sempre orientato ad offrire alle donne del nostro Paese reali strumenti reali strumenti di emancipazione nel difficile cammino verso la piena parità nelle opportunità di vita e di lavoro. Da un suo disegno di legge, ad esempio, ebbe origine la legge n. 215 del 1992, che favoriva per la prima volta azioni positive in favore della imprenditoria femminile. La Presidenza, aderendo alle proposte avanzate da numerose senatrici, ha avviato le procedure per la pubblicazione dei discorsi parlamentari della nostra illustre collega.

È difficile non sentire la responsabilità nel rendere onore alla nostra collega Alma Agata Cappiello. La sua vita è stata troppo breve, anche se di una ricchezza straordinaria, e questo ha reso meno accettato il suo commiato. Il presidente Giorgio Napolitano, nel marzo 2007, in un messaggio inviato in un incontro a lei dedicato a Milano, offre uno sguardo lucido sulla personalità di Alma: «Un percorso, quello della Cappiello, che ha preso le mosse dal Consiglio comunale di Milano e dalla militanza nelle file del Partito Socialista, ed è continuato nelle Aule parlamentari, dove l'ho conosciuta sempre impegnata nella promozione di un'effettiva parità tra uomo e donna; successivamente, in un tormentato passaggio di vita politica e anche personale, resta esemplare la fiera coerenza con cui ha vissuto anni difficili per il suo partito e la sua salute, e il coraggio con cui ha saputo guardare al futuro senza rinnegare il valore di una lunga esperienza politica». L'azione politica di Alma Agata Cappiello tocca i punti più salienti del riformismo italiano. In tutte le esperienze il suo è un procedere autonomo, proprio di una protagonista del riformismo socialista di cui, come ha detto Paolo Pillitteri in una dichiarazione l'8 novembre 2006, «lei rappresentò l'ala più sensibile ai cambiamenti e attenta ai bisogni nuovi che si manifestavano nella società». Questo giudizio di Pillitteri è tanto più vero laddove si affronti il contributo di Alma alla storia delle donne. È indubbiamente in relazione con il dibattito femminista che si svolge in Italia e nel mondo, ma il suo approccio, anche se di tale dibattito si nutre, non è mai un'applicazione ripetitiva, stanca e astratta di esso. Il suo è un modo di vedere le cose legato all'esperienza delle donne della sinistra italiana ed europea, del PSI, e alle donne laiche e cattoliche del centrosinistra, con le quali trae la responsabilità di Governo. L'assunzione di responsabilità è decisiva per Alma. Se quello in cui si crede è forte, allora deve poter cambiare le cose. La forza delle idee è anche forte responsabilità. In lei c'è un legame fortissimo tra etica della convinzione ed etica della responsabilità di weberiana memoria. Di Alma spesso le dirigenti socialiste, ma anche le donne provenienti da altri mondi, hanno messo in rilievo l'azione incessante per l'unità delle donne. Ebbene, questa unità non è possibile concepirla senza il convincimento, in Alma, che, per affermare i loro diritti, le donne debbano essere unite; e che l'unità è legata a questa ambizione: quella di cambiare le cose. Altrimenti, idee, anche giuste, rimangono semplici punti di vista. Tale impianto, il cui centro è costituito da un anello riformista, ha fatto sì che il dibattito intorno ai diritti, anche quando vivace, è sempre stato rispettoso delle diverse identità e tradizioni culturali e religiose. È questo suo modo di intendere la politica che la porta a una produzione molto ricca di progetti di legge e ad essere presente nel dibattito politico e culturale, oltre che a curare numerose pubblicazioni: una su tutte, il "Codice Donna". C'è un vero e propria asse nelle sue proposte: l'attenzione ai diritti civili non è mai contrapposta a temi considerati "più tradizionali", come quelli legati alla famiglia. Anzi, all'opposto, Alma Cappiello non solo non li vede in contraddizione, ma li colloca dentro una visione moderna, sia del *welfare* che dei rapporti tra le persone. Così, le proposte per la convivenza e le dieci proposte per sostenere le famiglie sono in entrambi i casi innovative e rispondenti ai bisogni reali dei cambiamenti intervenuti nella società italiana. Anche relativamente ad altri due temi, è il filo innovativo che unisce le proposte non si sofferma esclusivamente sulla violenza alle donne come elemento residuale e sulla violenza presunta ai minori, ma tematizza la dimensione sociale e familiare della violenza e l'aumento della violenza sui minori. Nel secondo caso, propone una legge sull'imprenditoria femminile e una sulle azioni positive. Quest'ultima è il frutto di un dibattito internazionale, ma l'innovazione portata dal testo non è di poca cosa, con l'introduzione dell'onere della prova nell'azione discriminatoria, dell'inversione proprio dell'onere della prova. Si potrebbe continuare, colleghe e colleghi, ma vorrei invece sottolineare di Alma un altro aspetto che attiene al suo modo di relazionarsi ad altre donne e alla responsabilità che ha sempre sentito nel lavoro politico con le donne. Per la senatrice Cappiello, nessuna nasce sola o, per meglio dire, è meglio non nascere da sola. Si ha bisogno anche di madri politiche o, comunque, si ha bisogno di riconoscere le altre, di stimarle: non per mera generosità, ma per la propria identità. Recentissime come soggetti sociali, le donne per essere più forti hanno bisogno di conoscere chi le ha precedute. Escluse per millenni dalla scena pubblica, hanno la necessità di vedere come le altre ci sono entrate, come hanno fatto, per trarre forza dalla loro esperienza. A questo si ascrive la sua attenzione alla storia, anche recente, delle donne. Lei ha avuto forti relazioni con le donne, anche di un'altra generazione. Una di loro è stata Elena Marinucci; a lei la presenta un amico importante del padre, Bettino Craxi, e all'inizio ne riceve la diffidenza, come la Marinucci ha dichiarato in un recente convegno, per poi diventarne, in poche ore, un'amica e una compagna indispensabile nella battaglia politica. Per un lungo periodo Alma non ha partecipato alla vita politica di nessun partito. Ha sofferto moltissimo la crisi del PSI seguita a Tangentopoli e al destino di Bettino Craxi e ha combattuto a testa alta perché un secolo di vita e di storia socialista non venissero ricondotte solo a vicende giudiziarie. Leale a Craxi e alla sua famiglia, partecipa fino alla fine alle vicende del dirigente socialista. Alma si apre, negli ultimi anni della sua vita, alla possibilità della costruzione di un nuovo soggetto riformista. Lo fa attraverso il gruppo dei Riformatori per l'Europa, cofondatori dei Democratici di Sinistra, in particolare attraverso Benvenuto e le sue amiche e colleghe, Franca Donaggio e Beatrice Magnolfi, ed entra, al congresso del 2004, nell'Assemblea nazionale. Nel chiedere l'iscrizione ai DS, porta con sé tutta la sua fierezza di dirigente socialista. Nella lettera a Piero Fassino, segretario dei DS, pubblicata su «l'Unità», si comprende bene la sua intatta passione e tensione nella richiesta richiesta di «una politica etica, una politica di valori, che si esprime attraverso un pluralismo di valori, quali la lealtà, le scelte responsabili, la ricchezza delle diversità, le politiche di pari opportunità, la solidarietà intesa come reciprocità tra pari». Ed in un altro passo motiva il perché della sua adesione ad un nuovo progetto politico nella volontà di dare «un apporto essenziale al cammino di unificazione del riformismo italiano». Un progetto - colleghe e colleghi - grande, ambizioso, a cui siamo ancora chiamati e il cui percorso ancora non è semplice e di cui lei, purtroppo, non ha potuto compiere che pochi passi. I due decenni che ci stanno alle spalle sono ancora poco indagati. L'antipolitica appare ancora, per una parte della classe dirigente e dei cittadini, la risposta più forte, in sintonia con la storia delle fragilità dello Stato italiano. Per la Cappiello la politica deve essere una forza autonoma e non subalterna a nessun altro potere. Con la stessa dignità ha immesso le sue radici particolari, napoletane, nella città di Milano, e nelle sue istituzioni, a partire dal Consiglio comunale, dove ha vissuto e dov'è stata riconosciuta come una delle sue figure più di spicco. Lasciatemi dire alla fine, colleghe e colleghi, ciò che Roberto Gervaso ha avuto modo di dire di Alma: dire di Alma: è «un magnete glassato». È una definizione che coglie la sua personalità. Bella, giovane, colta, professionista in ascesa nel mondo del diritto. Poteva permettersi di giocare molto di più sulla glassa. Invece, con il lavoro incessante, che non badava ad orari, come tutti raccontano, la glassa non era solo un modo per rendere più forte l'azione del magnete, ma pure la consapevolezza che la forza del magnete sta anche nel non rinunciare alla propria femminilità. Alma, una grande protagonista e, soprattutto, una riformista, che ha speso tutta la sua vita per gli ideali di libertà e giustizia, per rendere più moderno e forte il nostro Paese e per la dignità e i diritti delle donne.

Signor Presidente, onorevoli senatori, Alma Cappiello era una democratica, una socialista, una riformista, ma soprattutto una "donna in politica", che si è sempre battuta contro le discriminazioni di genere e per la libertà di accesso al mondo del lavoro. La sua attività parlamentare, passata nelle file del Partito Socialista di Bettino Craxi, è stata relativamente breve, ma da una forte intensità e partecipazione alle cause che le erano più care. Nei suoi dieci anni passati tra il Senato e la Camera, non ha mai ritenuto opportuno risparmiarsi o mettersi in retrovia: al contrario, è riuscita, con coraggio e senso critico, a lasciare un segno indelebile nella nostra società e nell'ambito di quelle che oggi, anche grazie alla sua sensibilità, definiamo «pari opportunità». Fu ispiratrice e, se vogliamo, anticipatrice di due leggi che hanno attualizzato e migliorato il nostro ordinamento: la n. 125 del 1991 (che affronta un tema ancora attuale, come quello dell'accesso delle donne nel mondo del lavoro) e la n. 215 del 1992 (che regola l'imprenditoria femminile). La sua attività politica, negli anni, si è concentrata anche sulle tematiche dell'adozione e dell'affido, argomenti che ancora oggi animano il dibattito sociale e politico e che devono farci riflettere su quanto, anche grazia ad Alma Cappiello, sia stato fatto e su quanto ancora si possa fare. Negli anni di Tangentopoli, al dolore per la scure

sposò la causa dei Democratici di Sinistra, cui non fece mancare fino all'ultimo momento il suo contributo critico e la sua vivacità intellettuale. Odiava la politica costruita sul trasformismo, sulle furbizie, sul vuoto dei contenuti; si è sempre battuta, al contrario, per una politica vera, concreta e più "femminilizzata", che doveva coincidere, secondo lei, nell'incrocio tra intelligenza e sentimenti. Molti, nel ricordarla, l'hanno definita una *pasionaria*: la sua vera passione erano i diritti delle donne, presto diventati una missione che ha caratterizzato tutto il suo percorso politico e di vita. grazie a donne come la Cappiello che temi, una volta considerati tabù per le donne, oggi sono diventati patrimonio comune e condiviso della nostra società.

Presidente, colleghe e colleghi, oggi ricordiamo una donna, Alma Cappiello, che ha lasciato sicuramente un segno nella vita politica del nostro Paese. Milanese, ma di famiglia napoletana, avvocato, socialista, si avvicinò alla politica con grande passione e grande naturalezza, facilitata in questo anche dall'ambiente familiare. Nel 1984 fu coordinatrice della Commissione nazionale per le pari opportunità, istituita per la prima volta dal Governo Craxi e presieduta da un'altra grande donna della politica italiana, Elena Marinucci; Commissione che pubblicò il primo "Codice donna", una raccolta di tutta la legislazione nazionale e internazionale vista dalla parte delle donne. Nel1985 venne eletta consigliere comunale a Milano, nel 1987 alla Camera dei deputati e nel 1994 al Senato. Ho incontrato Alma Cappiello una sola volta, quindi non posso dire - e me ne dispiace - di averla conosciuta bene. Ho cercato allora di ricostruire la sua figura attraverso il suo operato e basta analizzare il suo lavoro in Parlamento per capire di quale donna stiamo parlando. Era un'esperta di diritto e proprio all'implementazione dei diritti delle donne e dei bambini, delle fasce deboli in generale, ha indirizzato la maggior parte del suo lavoro.

Macredo che, per inquadrare in modo più completo il suo lavoro parlamentare, debbano essere anche ricordate altre proposte, come quella per la tutela della maternità delle lavoratrici autonome o quella sulle competenze dei tribunali per i minori e la famiglia, norme contro la violenza sessuale. Si occupò a lungo anche di affido e adozioni e nel 1988, cioè vent'anni fa, cercò anche di affrontare il problema delle nuove convenienze; tema difficile e tuttora molto controverso. Come ho già ricordato, molte delle sue proposte sono diventate legge dello Stato e anche da questo si può comprendere come riuscisse a coagulare attorno a sé un consenso che andava ben al di là dell'appartenenza politica, oltre l'ideologia, sempre dritta al risultato, sempre nel merito dei problemi. Una donna capace di dialogare alla pari anche con donne che appartenevano ad altre culture politiche, convinta che una maggiore partecipazione femminile avrebbe portato linfa vitale alla società e alla politica italiana. Amava definirsi una socialista riformista e sicuramente, grazie anche al suo appassionato lavoro, ha contribuito a valorizzare un'intera generazione di donne che stanno diventando, anche se con molta fatica, classe dirigente di questo Paese. Molto provata dalle vicende che travolsero il Partito socialista nella bufera di Tangentopoli, in un clima di forsennato e generico giustizialismo che cancellò di fatto il Partito socialista dal panorama politico italiano, aderì dopo alcuni anni ai Democratici di Sinistra che però - questo è il giudizio di Elena Marinucci - non le diedero il ruolo che meritava; ma - come ha detto sempre la Marinucci - quando la propria casa brucia e la passione politica è tanta, se ne cerca un'altra. Ho letto che una delle sue frasi ricorrenti era: "Riprendiamoci la politica". Sinceramente non so esattamente cosa volesse dire. Mi piace però pensare che volesse dire: "Torniamo a fare politica per cercare di risolvere i problemi delle persone", che in sostanza è l'unico vero motivo che dovrebbe spingere tutti noi a fare politica. *(Generali

davvero per aver voluto ricordare quest'anno, a due anni dalla scomparsa, quando piangevamo la prematura scomparsa di Alma Cappiello, il suo straordinario personaggio, Una difficilissima sintesi politica, quella compiuta da Alma e dalle donne della sua generazione, come la sua, senatrice Serafini, che dovevate traguardare il Paese dall'essere un Paese in via di sviluppo al divenire finalmente un Paese moderno. Una sintesi giocata sul crinale, spesso delicato, dei discrimini dei diritti civili, antichi e moderni, e della discriminazione, vecchia e nuova, che impediva l'avanzamento della condizione femminile. che ho avuto la fortuna di essere formata nel solco del suo lavoro di responsabile delle donne socialiste e che ho avuto la straordinaria fortuna di essere testimone della sua incessante attività tra partito e Parlamento, associazionismo e società politica, io, figlia sua, come lei lo era di Elena Marinucci, è come se la vedessi qua, oggi, in quest'Aula, instancabile nell'essere donna e politica a tutto tondo. Quella politica non subalterna a nessuno, riformista sempre, in ogni atto politico, pervasa di quell'anticomunismo che affonda le radici nell'autonomismo e nella socialdemocrazia, della quale lei era moderna testimone fin dagli inizi della sua carriera, da quando nelle istituzioni era consigliere comunale a Milano, nel 1985, al fianco di Bettino Craxi, in quella Milano da qualche stolto definita "da bere" che lei, senatore Veronesi, sono certa ricorderà in qualità di testimone e di protagonista di quegli anni; e poi deputata, responsabile della Commissione nazionale per la parità, istituita per la prima volta nel nostro Paese sotto la Presidenza del Consiglio di Bettino Craxi e, soprattutto, dirigente nazionale Grazie. Ella chiude un filo di perle lungo cento anni di socialismo riformista, che ha visto brillare figure fulgide come Anna Kulishov, teorica del riformismo e madre della prima legge di tutela della maternità, come Argentina Altobelli, prima segretaria del sindacato dei braccianti (allora il più potente), come Anna Maria Mozzoni, fondatrice dei primi asili nido sui luoghi di lavoro in quella Milano culla del riformismo, e come Lina Merlin, che mise fine al commercio di carne umana legalizzata nelle case chiuse. Questa è la fonte alla quale si abbeverò Alma Cappiello, che raccolse e trasferì poi in tutti i suoi atti parlamentari, in tutti i suoi numerosissimi disegni di legge, uno tra tutti, anticipatore di tanti altri, quello sulla disciplina delle famiglie di fatto, ma anche quello dei congedi parentali, dell'assegno e del sostegno alla maternità, della tutela dei minori, della tutela dei minori, quelli in materia di asili nido, di infortuni delle casalinghe e di istituzione dei consultori familiari. Tutto questo racchiuso in una grande opera di giurisprudenza che altre colleghe hanno citato, che è quel famoso "Codice Donna" che porta per tutti noi il suo nome. Cento anni di socialismo conclusi nell'ultima responsabile femminile, lei, Alma Cappiello, che dovette penare molti anni, insieme con tante di voi, per vedere approvata dal Parlamento italiano la legge contro la violenza sessuale che prima di allora, come tutti noi ricordiamo, non era violenza contro la persona. Quel famoso soffitto di cristallo, contro il quale noi ancora oggi combattiamo e che lei combatteva più di tutti gli altri, non è ancora stato infranto e non tutti i diritti di cittadinanza, ancorché scritti sulla carta, si sono ancora compiutamente realizzati. Ma non l'ha vinta l'ingiustizia politica di vedere finire con lei la storia del Partito socialista italiano: l'ha vinta, invece, quel male tremendo che l'ha piegata fino alla morte. Ma fino all'ultimo è rimasta vicino alle lotte, anche le più moderne, delle donne italiane, per ribadire, conquistare e riconquistare ogni giorno pezzi di libertà e di dignità. Oggi certamente il suo pensiero sarebbe rivolto, così come in tanti di noi, a quelle donne, a quelle che lei simpaticamente chiamava, chiamando ciascuna di noi, "piccole", piccole sorelle che girano per le nostre strade, nella sua Milano in particolare, con il capo coperto in virtù di una legge assurda che qualcuno assimila al Corano, ma che, in realtà, è solo un arcaico e quanto mai ottuso modo di intendere la diversità tra uomini e donne, piegando le donne sotto il calcagno di una follia che si chiama integralismo islamico. Quella oggi sarebbe la sua battaglia. Ecco perché il nostro pensiero va ad Alma Cappiello, alla sua straordinaria figura politica e alle contaminazioni che, insieme con molte parlamentari di tanti schieramenti politici e colleghe del suo tempo, è riuscita a svolgere nelle diverse aree politiche, nelle diverse aree del Paese, nelle trasformazioni della nostra società. Ecco perché le senatrici e i senatori di Forza Italia, con tanti socialisti veri, oggi la piangono e la ricordano sempre stringere tra le mani il suo garofano.

Ricordo innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, in seconda lettura si procede unicamente all'accertamento preliminare della conformità della copertura del disegno di legge finanziaria alle regole stabilite in questa materia dalla vigente legislazione contabile. Ciò premesso, sentito il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato e preso atto anche della posizione assunta in materia dal Governo, comunico le determinazioni della Presidenza, che prego il senatore Segretario di leggere all'Assemblea.

si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge finanziaria in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato recante lo schema di copertura nella versione approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura del disegno di legge finanziaria 2009 sono costituite da nuove o maggiori entrate dell'articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nell'articolato che disposte dalla tabella E - per il solo 2009

quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sul DPEF per il 2009-2013 tenuto conto della relativa Nota di aggiornamento (articolo 11, comma 6, della legge n. 468, modificata), si rileva che il vincolo del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è rispettato per il primo anno (2009) ricompreso nel triennio del bilancio pluriennale: esso risulta infatti coincidente con l'obiettivo fissato nella predetta Nota ed è pari a 33,6 miliardi. Per il 2010 e 2011 la Nota di aggiornamento indica solo i valori programmatici, identici a quelli di cui all'articolo 1, comma 2 del disegno di legge finanziaria. I saldi a legislazione vigente per il 2010 e 2011 risultano invece più elevati di quelli programmatici esposti da ultimo nella Nota di aggiornamento. Al riguardo, si prende atto dell'impegno del Governo ad attivare ulteriori misure di razionalizzazione tali da rendere possibile l'avvicinamento tra il saldo netto da finanziare a legislazione vigente ed il corrispondente valore programmatico per ciascuno dei due anni indicati. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2009-2011, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate e dal rispetto degli obiettivi di fabbisogno di cassa del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Le varie norme di cui al disegno di legge finanziaria forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2009. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggioramento dei valori di correzione associati al disegno di legge finanziaria in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di fabbisogno del settore statale e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 5 e 6 del richiamato articolo 11 della legge n. 468 modificata». finestra"). Comunico che sono deferiti alla 5a Commissione permanente, in sede referente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali, disegni di legge nn. 1209 (Legge finanziaria per l'anno 2009) e 1210 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011).

Signor Presidente, voglio sottoporle un problema che riguarda l'ordine dei lavori, ma che è anche un richiamo al nostro Regolamento.

Abbiamo più volte denunciato, in questi mesi, il fatto che il Parlamento si occupi pressoché totalmente di decreti-legge; ne hanno parlato il presidente Zanda e altri colleghi in altre sedute: 30 decreti-legge dall'inizio della legislatura. Ne rimangono, ad oggi,

il fatto che assistiamo - è avvenuto già per gli altri decreti, ma rischia di avvenire in misura particolare per quello che stiamo esaminando - ad una dilatazione del contenuto del provvedimento legislativo di conversione, che rischia di assumere, per come si presentano i testi degli emendamenti, il carattere dell'abnormità. Le chiediamo, quindi, signor Presidente, di valutare attentamente i criteri di ammissibilità richiamando in particolare il contenuto degli articoli 78 e 97 del nostro Regolamento, dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, della prassi e dei precedenti, anche giurisprudenziali, che si sono espressi

all'articolo 97, comma 1, sancisce l'improponibilità degli emendamenti e delle proposte estranei all'oggetto della discussione, con una formulazione quindi un po' più ampia.

l'interpretazione che è stata data delle norme regolamentari cui ho fatto riferimento, in particolare dell'articolo 97, comma 1, ci consente di avere un quadro sufficientemente chiaro, che va quindi ben adattato al provvedimento che stiamo esaminando. In particolare, voglio richiamare una circolare presidenziale che, al punto 5.1, prevede che l'articolo 97, comma 1, del Regolamento va interpretato nel senso che debba essere dichiarata l'estraneità all'oggetto della discussione degli emendamenti, non solo ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in senso stretto, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione; in questo caso dell'Aula. Ricordo anche che, nel 2002, l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nel rinviare alle Camere

nel censurare l'aggiunta di norme che esulavano dal contenuto proprio del decreto, ebbe a dire che quel modo di procedere configura uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge, non conforme, e leggo testualmente, signor Presidente: «al principio consacrato nell'articolo 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale, in quanto preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza, e deve quindi essere del pari rigorosamente osservata. Tutto ciò» diceva il presidente Ciampi «mette in evidenza la necessità che il Governo, non soltanto segua criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge, ma vigili successivamente, nella fase dell'esame parlamentare, allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali La Corte costituzionale si è conformata a questi principi, nel senso che con due recenti sentenze, che lei certamente conosce, la n. 171 del 2007 e la n. 128 del 2008, ha ribadito il principio dell'inammissibilità di norme estranee alle materie disciplinate dal decreto-legge il rischio, nel censurare provvedimenti di conversione di decreti-legge, dello stravolgimento del procedimento legislativo in contrasto con le previsioni dell'articolo 77 della Costituzione, anche in rapporto

di impresa in amministrazione straordinaria, con tutte le conseguenze in ordine al diritto dei lavoratori, in quanto legata alla materia della cessione di azienda. Vi è poi addirittura una norma di interpretazione autentica, un emendamento presentato dal Governo, in materia di fornitura di energia elettrica, che non ha nulla a che fare con il contenuto di questo decreto; un'altro emendamento riguarda la collaborazione del Ministero delle infrastrutture con la BEI per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, che non c'entra niente con questo provvedimento e che non presenta certamente i caratteri dell'urgenza; un altro ancora riguarda i programmi nazionali "Urban Italia" che non ha nulla a che vedere con il contenuto di questo decreto e che non presenta certamente i caratteri dell'urgenza. Vi erano norme molto gravi, che riguardavano la costituzione della società Difesa Servizi, la valorizzazione degli immobili della Difesa,

È rimasto invece - questi che ho citato da ultimo sono emendamenti ritirati e mi auguro che a nessuno venga in mente di ripresentarli in Aula - il differimento di termini della disciplina dell'arbitrato, come era stata formulata in occasione della legge finanziaria dello scorso anno. anno. Signor Presidente, io credo che lei debba fare un lavoro che rispetti questi principi costituzionali, regolamentari, giurisprudenziali, di prassi parlamentare, conto anche di un altro aspetto, di cui parlerà tra poco il senatore Morando, che riguarda i profili di onerosità in rapporto alle regole che governano la sessione di bilancio che lei ha aperto poc'anzi. chiediamo, quindi, formalmente di dichiarare inammissibili o improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, tutti gli emendamenti che presentano le caratteristiche a cui

che durante la sessione di bilancio, che si apre con le comunicazioni che ella ha testé rivolto all'Assemblea del Senato, vengano discussi e soprattutto approvati provvedimenti di legge che hanno carattere oneroso, cioè che incidono sul bilancio dello Stato. Ovviamente, questa norma regolamentare prevede - dico ovviamente perché era naturale che così fosse - un'eccezione: durante la sessione di bilancio non si possono discutere disegni di legge che implichino oneri per la finanza pubblica, sia in termini di minori entrate sia in termini di maggiori spese, all'unica condizione che non si tratti di disegni di legge di conversione di decreti. Qual è la *ratio*, signor Presidente, colleghi, di questa regola e della sua eccezione? La *ratio* della regola è prestissimo spiegata: tutta la sessione e tutta la decisione di bilancio è fondata sulla predisposizione del documento che viene definito "bilancio a legislazione vigente". È del tutto evidente che se durante tale sessione i dati i dati del bilancio a legislazione vigente vengono modificati da innovazioni della legislazione vigente che implicano oneri ciò vanifica la base la base della decisione di bilancio. Ecco perché il Regolamento, molto opportunamente, prevede che, una volta aperta la sessione di bilancio, non è possibile, né discutere, né approvare disegni di legge che modifichino il bilancio a legislazione vigente. Naturalmente, la ragione dell'eccezione è altrettanto chiara: un decreto-legge è immediatamente in vigore, pertanto il decreto entra nella legislazione vigente. Quindi, il bilancio a legislazione vigente registra l'emanazione di un decreto secondo le norme e, di conseguenza, si considererà che il bilancio a legislazione vigente posto alla base della decisione di bilancio incorpori gli effetti finanziari determinati dall'approvazione del decreto. D'altra parte, l'approvazione di decreti è sottoposta a determinati vincoli, l'urgenza e così via, e quindi si sa che il Governo durante la sessione di bilancio non mettere in discussione il principio generale: durante la sessione di bilancio il Parlamento non può approvare leggi che, modificando la legislazione vigente di spesa o di entrata, modifichino di fatto il contenuto del documento fondamentale alla base della decisione di bilancio stessa.

se questa è la base razionale del nostro Regolamento, non possiamo, e a mio giudizio lei, signor Presidente, ed i Presidenti di Commissione tutti non possono non apprezzare che si sta determinando un fenomeno particolarmente insidioso per il rispetto di questa parte del nostro Regolamento. Cosa accade, signor Presidente? Che se il sottoscritto, o qualsiasi altro senatore, presentasse domani mattina un disegno di legge che consta di cinque articoli, tutti onerosi, o che comunque incidono sul bilancio a legislazione vigente, e ci fossero le condizioni e l'accordo per una sua discussione, tale disegno di legge non potrebbe essere ammesso da oggi pomeriggio in avanti alla discussione perché il nostro Regolamento lo vieta. lo stesso senatore o gli stessi senatori proponenti prendessero i cinque articoli di questo disegno di legge, ciascuno dei quali è oneroso, decidessero di presentare ognuno di quei cinque articoli onerosi come emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge, se non intervenisse una decisione circa l'ammissibilità, avremmo un evidente aggiramento della norma del nostro Regolamento. Infatti, alla fine, quegli emendamenti sarebbero tutti ammissibili e durante la sessione del bilancio il Parlamento, il Senato in questo caso, si troverebbe ad approvare di fatto un disegno di legge che, a forza di Regolamento, non avrebbe dovuto essere ammesso alla discussione, sia pure approvato, come si direbbe nel nostro gergo, per parti separate.

della legge finanziaria in vigore ed hanno valore per il 2009, 2010 e 2011, incidendo direttamente sulla tabella C della legge finanziaria che noi dobbiamo discutere e alla fine approvare;

la Commissione bilancio, poiché questi emendamenti dalle Commissioni di merito vengono considerati ammissibili, si trova nella seguente situazione: comincia la sessione di bilancio, con la relazione sulla finanziaria e ha ricevuto un documento (legge finanziaria e legge di bilancio) approvato dalla Camera dei deputati;

la tabella C della legge finanziaria tiene conto degli effetti finanziari dei decreti-legge in corso, ad

Il vero problema è che qui stiamo parlando di iniziative parlamentari, signor Presidente. La Commissione bilancio - credo che il presidente Azzollini non avrà difficoltà a convenire con me - si trova in un fortissimo da un lato, abbiamo un emendamento che coprendosi, ad esempio, con un taglio lineare della tabella C, se lo esaminassimo a prescindere dal fatto che siamo in sessione di bilancio, non meriterebbe parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. meritare parere contrario senza riferimento all'articolo 81 perché la tabella C non è una vacca da mungere (mi perdoni l'espressione un po' volgare), ma è una tabella che è è uniformata, nelle sue dimensioni, a coprire la legislazione vigente: ma dal punto di vista formale, l'emendamento è non colpibile con un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con tutte le conseguenze che questo determina. Se però la Commissione bilancio esprime parere favorevole su quell'emendamento, dopo qualche minuto si trova ad esaminare una legge finanziaria che non ha più in tabella C la cifra che c'è scritta nella legge finanziaria, ma un'altra risultante dalla sottrazione tra quello che c'è scritto nella legge finanziaria e l'onere recato dall'emendamento su cui si è dato parere di nulla osta. Il risultato, signor Presidente, è che in Commissione bilancio non sappiamo cosa fare; normalmente potremmo dire potremmo dire una cosa che un tempo si diceva, e cioè che la Commissione bilancio dà parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo che l'approvazione di tale emendamento sia successiva all'approvazione della legge finanziaria. Ma lei capisce, signor Presidente, che in questo modo incorreremmo in una contraddizione irrisolvibile: possiamo discutere i decreti, perché sono decreti e non sono disegni di legge, durante la sessione di bilancio, ma poi, esaminando un emendamento al decreto-legge, diciamo che quell'emendamento si potrà votare soltanto dopo che avremo approvato la legge finanziaria, con il risultato di determinare il caos nei lavori del Senato, sia nelle Commissioni permanenti che in Aula.

La mia modestissima opinione, signor Presidente - mi rivolgo a lei perché faccia una valutazione equanime di quello che le sto dicendo; è del tutto evidente che non vi è alcuna intenzione ostruzionistica nel proposito che sto manifestando il Presidente del Senato e i Presidenti di Commissione, quando stabiliscono che l'emendamento ha queste caratteristiche, lo conferiscono alla Commissione bilancio solo per la verifica della possibile incidenza sul bilancio a legislazione vigente e, quando la Commissione bilancio ne verifichi l'incidenza, automaticamente lo dichiarano inammissibile - soluzione che considero perfettamente coerente con la lettera del nostro Regolamento - oppure

deferire immediatamente la questione alla Giunta per il Regolamento affinché possa esprimere un orientamento per la soluzione di una contraddizione che, in questo momento, mi pare assolutamente evidente. Per quello che vale,

della sua posizione circa la corretta copertura della legge finanziaria, ha ammesso che una gestione dell'ammissibilità che renda compatibile,

alcune osservazioni di merito, politico ed economico, che le questioni poste ci costringono a dover affrontare. La prima di esse la quantità dei tagli lineari fatti, che incidono non soltanto sulla tabella C, ma anche, ad esempio, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica o sul Fondo per le aree sottoutilizzate o sui fondi del Ministero degli affari

e delle istituzioni di quelle tabelle o di quei fondi. Più precisamente, l'insieme degli emendamenti che nella legge finanziaria sono assoggettati ad una compensazione e che nei decreti-legge, in particolare quelli non collegati alla finanziaria, non sono assoggettati a compensazione, ma soltanto a copertura, costringono la Commissione bilancio a dover dare un parere teoricamente compatibile con l'articolo 81, quarto comma, ma che nel merito potrebbe compromettere

La questione si complica ulteriormente perché per la maggior parte di questi provvedimenti vale un'altra ipotesi di censura: spesso utilizzano fondi di parte capitale per fondi di spesa corrente. Ciò vale per la tabella C, dove ci sono fondi di parte capitale e certamente per il Fondo per le aree sottoutilizzate. Naturalmente, questo questo degrada la qualità del bilancio, perché è ben noto che l'utilizzo di fondi in conto capitale per il finanziamento di spese correnti degrada i fondi di parte

si capisce che la degradazione è notevolissima e impedisce spese per investimenti in maniera tripla rispetto alla spesa corrente che si finanzia. Chiaramente, tutto questo ha effetti notevoli. notevoli. La Commissione bilancio, in linea di prassi, si sta comportando seguendo una rigorosissima interpretazione dell'articolo 81,

perseguire le scelte di politica economica effettuate all'interno del bilancio dello Stato e discusse in Parlamento, scelte che ci vedono su posizioni diverse, ma che nessuno ritiene di poter compromettere, tanto meno la maggioranza.

cui abbiamo dato un parere sul prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria, che lei è tenuto ad asseverare con la sua propria responsabilità e che presenta anche i suddetti problemi, non con specifico riferimento al prospetto di copertura (che infatti non li pone), ma con con una rilevanza su aspetti procedimentali, formali di bilancio e sostanziali di politica economica, che abbiamo ritenuto necessario rilevare. Anche per questo, signor Presidente, non so se abbiamo fatto bene, ma

non avendo concluso con questo unico emendamento, ma ci sembra assolutamente rilevante per il nostro lavoro e di ciò la ringraziamo.

un'eccezione che verte sulla inammissibilità per materia degli emendamenti; il senatore Morando ha sviluppato un altro tipo di osservazione acuta sulla

un compiuto approfondimento delle osservazioni dei colleghi perché le ritiene significative e interessanti, sicuramente dotate di un *fumus* che merita un'attenta analisi. Verificheremo anche i precedenti, ma non ci faremo soltanto condizionare da questi; svolgeremo un'attenta analisi e questo assicuro all'Aula.

poter avere le idee più chiare e poter assumere delle decisioni, non escludendo anche l'ipotesi di una convocazione della Giunta per il Regolamento. La Presidenza, però, intende prendersi il doveroso e opportuno spazio temporale per poter riflettere. condividete questo percorso, io procederei in siffatta maniera.

Dirò, anche per osservare quello che è stato il comportamento della Commissione di merito Grazie. a un rigore assoluto di rispetto dei deliberati della Commissione bilancio, nel senso di non aver approvato nessun emendamento che avesse il parere contrario della Commissione bilancio. Anche nel merito, doverosamente accoglienza agli emendamenti proposti dai colleghi, ha con rigore tenuto una condotta abbastanza lineare in ordine all'ammissibilità degli emendamenti più rilevanti, ottenendo il ritiro dell'emendamento relativo all'arbitrato e ottenendo altresì il ritiro dell'emendamento del Governo in ordine alla società detto per non togliere alle Commissioni di merito il giusto spazio di dibattito. Detto questo, farò una breve illustrazione sul complesso delle norme che questo disegno di legge contiene.

contiene una norma, afferente soltanto all'anno 2008, di revisione dei prezzi negli appalti dei lavori pubblici. dei lavori, anche per effetto dello straordinario incremento del prezzo delle materie prime, in particolare dei prodotti petroliferi, e di conseguenza di alcuni materiali di costruzione ad essi collegati,

l'aumento straordinario dell'acciaio (che è arrivato ad incrementi del 150 per cento) e del rame, solo per fare alcuni esempi. È chiaro che in moltissime situazioni si è determinato il blocco

settori cioè in cui l'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi è stato particolarmente influente.

e che con questo provvedimento vengono riportati all'interno del bilancio dello Stato e destinati ai suddetti fini.

si riferisce al G8 della Maddalena e prevede fondi per complessivi 233 milioni di euro, la metà circa dei quali (cioè 122 milioni 122 milioni di euro) viene reperita all'interno di delibere CIPE già approvate che utilizzano fondi FAS destinati alla tratta, quindi, di opere previste all'interno della programmazione 2000-2006. Altre risorse (pari a 111 milioni di euro) sono relative alla programmazione 2007-2013, sempre riferita ai fondi FAS e ai rapporti con la Regione Sardegna. I commi da 2 a 5, invece, si riferiscono all'attuazione di un provvedimento già assunto dal precedente Governo, che riguarda la regolazione della restituzione del vantaggio che, a valle del terremoto, venne riconosciuto agli enti pubblici e privati di Umbria e Marche, quando venne sospesa l'obbligatorietà di versare i contributi previdenziali per i soggetti pubblici e privati che risiedessero o operassero all'interno di queste Regioni nelle aree colpite dal terremoto.

le regole che disciplinano la restituzione del 40 per cento delle somme non versate per effetto delle ordinanze emesse a valle del terremoto. Nel corso dell'esame del provvedimento sono stati presentati due emendamenti da parte del Governo. Il primo riguarda un'interpretazione autentica delle modalità del cosiddetto *décalage* e quindi della diminuzione del prezzo dell'energia riferito a determinati soggetti utilizzatori

emendamento presentato dal Governo riguarda l'inapplicabilità delle norme dell'articolo 2112 del codice civile nei casi in cui

non c'entrerebbe nulla). Quindi, nel caso di aziende in amministrazione straordinaria, in caso di vendita di *asset* parziali, quindi di rami d'azienda, non è applicabile l'articolo 2112 del codice civile. Questo è l'aspetto normativo che regola l'emendamento del Governo presentato all'interno del provvedimento.

consistenza perché era relativa a finanziamenti per un miliardo e 440 milioni per l'anno 2009 e dello stesso ordine per gli anni successivi, successivi, relativa ai contratti di programma e ai contratti di servizio per le Ferrovie dello Stato, è stata ritirata dal Governo stesso, consentendo quindi un dibattito al di fuori di questo provvedimento relativo all'utilizzo dei fondi FAS. riguardo, c'era un emendamento di un collega relativo ad una parte di quell'emendamento del Governo,

Sono stati acquisiti i pareri di merito - tutti favorevoli - della Commissione affari costituzionali, della Commissione bicamerale per gli affari regionali, della Commissione finanze, della Commissione agricoltura,

recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, è volto, secondo la Relazione tecnica presentata dal Governo, sia ad emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, sia a promuovere lo sviluppo economico con specifico riguardo al mantenimento dei dei livelli di competitività nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, sia a far fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni Comuni

in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. La rubrica dell'articolo 3 del provvedimento in oggetto, recante interventi in materia di protezione civile, evoca impropriamente la materia della protezione civile, anche se autorizza una spesa per la Presidenza italiana del G8 di ben 233 milioni di euro. Il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 1 incrementa il fondo di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazione contabile con le autonomie locali, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011. Tale incremento viene effettuato contestualmente all'istituzione di un fondo per l'adeguamento prezzi in materia di costruzioni, ma riguarda una disposizione contenuta in un decreto-legge

Al riguardo si osserva che né nella motivazione del decreto-legge, né nell'articolato, né nella relazione governativa si spiega la ragione dell'intervento normativo di cui al terzo periodo dell'articolo 1, sebbene la Corte costituzionale, con sentenza n. 128 del 2008, abbia dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni del decreto-legge n. Ribadendo in tale occasione i principi enunciati dalla precedente sentenza n. 171 del 2007, relativamente alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza delle disposizioni contenute nei decreti-legge, la Corte ha stabilito che l'esistenza di tali requisiti non può essere sostenuta da una mera ed apodittica enunciazione, ma deve trovare puntuale spiegazione nella motivazione del decreto-legge. Una situazione analoga a quella relativa al terzo periodo del comma 11 dell'articolo 1 è riscontrabile anche all'articolo 3, comma 2, del provvedimento in oggetto, dove si interviene per la seconda volta su di una norma contenuta in un decreto-legge in corso di conversione da parte del Parlamento. Anche in questo caso non appare evidente la *ratio* dell'incremento finanziario, né la sua eventuale giustificazione con ragioni di copertura finanziaria e la Relazione tecnica del Governo omette di fornire indicazioni al riguardo. L'articolo 2 del provvedimento, recante norme relative ad interventi di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, non contiene disposizioni aventi carattere di urgenza, realtà, rivestono semmai natura esclusivamente procedimentale, poiché la concreta individuazione di strumenti normativi da utilizzare a sostegno dei settori in crisi richiamati dalla normativa viene demandata ad appositi decreti interministeriali. considerato che il decreto-legge è un atto con forza di legge che può essere adottato dal Consiglio dei ministri solo in casi straordinari di necessità ed urgenza; la straordinarietà di tale strumento normativo si riconduce alla deroga al principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento, sia pure per un periodo di tempo limitato (60 giorni), l'esercizio della funzione legislativa.

la necessità e l'urgenza e nel 2007, con la già citata sentenza n. 171, ha per la prima volta annullato un decreto-legge per carenza evidente dei presupposti e ha chiarito che la conversione parlamentare non può salvare il vizio, che incide sulla separazione dei poteri e non esclusivamente sul rapporto politico fra Parlamento e Governo. Considerato ancora che sussiste indubbiamente la necessità e l'urgenza di un intervento volto a risolvere la gravissima crisi infrastrutturale del Paese, a tale urgenza noi riteniamo si dovrebbe rispondere attraverso l'adozione di provvedimenti organici e strutturali nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, il provvedimento in oggetto costituisce l'ennesima dimostrazione di come quella infrastrutturale, cari colleghi della maggioranza, non sia affatto una priorità per l'agenda politica dell'attuale Governo, perché il testo in esame non prevede alcun finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di infrastrutture nel nostro Paese e dispone, anzi, pesanti decurtazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), senza chiarire se tali decurtazioni siano suscettibili di pregiudicare il completamento di interventi già avviati. Inoltre, il Governo ha previsto nel disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. una riduzione delle risorse destinate a nuove infrastrutture per il 2009, pari al 14,2 per cento in meno in termini reali rispetto all'anno 2008, considerato che la riduzione di tali risorse non fa altro che interrompere quel processo di recupero del livello degli stanziamenti attuato nelle due precedenti manovre di finanza pubblica del Governo Prodi (un incremento del 22,2 per cento nel 2007

apre una nuova finestra"). Ricordo che nella discussione sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

tocca diversi - e dobbiamo anche ricordare che il Parlamento e il decreto-legge non nascono oggi. Nella scorsa legislatura abbiamo molto più ampi e molto più eterogenei. Citerò soltanto come esempio, perché non fu un'eccezione ma fu, anzi, il paradigma della decretazione della scorsa legislatura, decreto Bersani, che toccava praticamente ogni argomento dello scibile umano. E ricordo che era un decreto-legge.

Grazie.

di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché finalizzato al finanziamento delle opere per il G8 e alla definizione degli adempimenti tributari per le Regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, si compone - com'è stato illustrato dal relatore - di tre articoli che disciplinano ambiti tra loro molto differenti, accomunati soltanto dal carattere di urgenza e straordinarietà per la crisi economica in atto. E qui occorre fare subito due rilievi. Il primo riguarda, innanzitutto, il carattere straordinario e contingente di un provvedimento il cui obiettivo principale avrebbe voluto essere quello di attenuare i significativi effetti che la crisi finanziaria internazionale sta cominciando a far sentire nell'economia reale, ma che nei fatti non coglie, risultando disomogeneo e privo di organicità. Di fatto, con l'iniziale presentazione di 35 emendamenti da parte della maggioranza e del Governo, ognuno diverso dall'altro e ognuno recante al suo interno vere e proprie norme nei più svariati ambiti di intervento (dalla difesa ai trasporti e alle infrastrutture, dalle concessioni ai contenziosi e alla deregolamentazione dei controlli), la maggioranza ha di fatto creato - e ancor più voleva creare - un decreto *omnibus*, di cui tutto si può dire, meno che abbia quei caratteri di urgenza e di straordinarietà che dovrebbero avere i decreti, per i quali viene richiesta la promulgazione del Presidente della Repubblica e sui quali il Parlamento è chiamato a convalidare la ratifica entro 60 giorni. Ancora una volta, la conversione di un decreto-legge ha fornito l'occasione per un vero e proprio assalto alla diligenza, snaturando la funzione stessa conferita alla decretazione d'urgenza. Tutto ciò, com'è stato detto anche da chi mi ha preceduto, è francamente inammissibile, sia sul piano del diritto, sia su quello della correttezza politica. Vorrei essere chiaro. Nessuno qui presente contesta le vostre prerogative di sostegno all'esercizio dell'azione di Governo: il punto è che devono essere esercitate nel pieno rispetto delle regole e della prassi costituzionale consolidata. È evidente invece che è in atto da tempo il tentativo da parte vostra di coartare consuetudini e rispetto istituzionale. Il secondo rilievo è nel merito del provvedimento che, come detto, non affronta in termini organici ed omogenei aspetti che, pur essendo condivisibili, sono tra loro talmente scollegati da renderlo inadeguato e di certo insufficiente a rispondere in maniera efficace agli obiettivi che in partenza si proponeva. È stato formato un *puzzle*, i cui pezzi non sempre si incastrano ed in Commissione è stato evitato persino il peggio; insieme, questi pezzi hanno concorso a creare un ginepraio di intendimenti che nulla o poco hanno a che fare con un progetto di sostegno a comparti maggiormente colpiti ed esposti alla crisi. Durante le audizioni in Commissione va tuttavia evidenziato che è emersa una sostanziale e per certi aspetti anche singolare identità di vedute tra le rappresentanze imprenditoriali e sociali, sia nell'analisi della sfavorevole congiuntura economica, sia nel merito del provvedimento. Questo come evidente conseguenza di una situazione che lascia pochi spazi di manovra ad elucubrazioni di tipo ermeneutico e che esige invece assunzione di responsabilità e piena finalizzazione delle risorse e degli interventi nell'interesse generale del Paese. Ma un aspetto sopra ogni altro non possiamo e non dobbiamo lasciar cadere: durante le audizioni è emersa unanime, con forza, come un grido di allarme, la necessità di intensificare la lotta alla criminalità organizzata che proprio negli appalti pubblici in alcune Regioni del nostro Paese trova non solo linfa vitale di alimento, ma anche il sostegno al proprio controllo del territorio e a forme sconsiderate di controllo ed oppressione sociale. Raccapricciante è stata la denuncia di frode di identità sporta dai rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori, consapevoli che essa costituisce il principale crimine contro il giusto profitto, contro la concorrenza e soprattutto contro i sacrosanti diritti dei lavoratori. Dalle loro denunce è emerso un affresco inquietante di un Paese in cui la legalità costituisce purtroppo un *optional* e che spesso non vede traduzione in certi contesti neppure nelle buste paga dei lavoratori. Al riguardo abbiamo presentato un ordine del giorno, accolto anche dalla maggioranza; ne abbiamo - voglio dirlo - apprezzato il gesto come le firme che si sono aggiunte.

Il tema, come sappiamo, riveste in questo momento particolare delicatezza in quanto interessa i costi di alcuni materiali da costruzione, le cui variazioni hanno inciso in modo considerevole nei rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti ed imprese esecutrici e, quindi, sulle possibilità di blocco di alcuni significativi cantieri necessari allo sviluppo del Paese. Eppure, possiamo dire senza il timore di essere smentiti, che il provvedimento è sicuramente insufficiente e inadeguato. Lo dico in una parola, non ha né una storia né un futuro. Non ricostruisce infatti la sede storica recente delle variazioni di prezzo dei materiali e soprattutto non dà alcuna certezza per le eventuali future oscillazioni che, se saranno ampie, potranno prefigurare davvero per molti cantieri il rischio della chiusura. All'articolo 2 il testo affronta il tema del recupero della competitività del nostro Paese in settori che hanno subito l'impatto dello *shock* dei costi dei prodotti petroliferi, *in primis* l'agricoltura, la pesca e l'autotrasporto. Il provvedimento affronta - ed ovviamente non risolve le criticità che si sono manifestate e che sono ancora in atto, preoccupandosi unicamente di distribuire a pioggia un po' di risorse, assolutamente insufficienti, destinandole qua e là senza alcun serio criterio di selezione. Sono insomma pannicelli caldi, impacchi che alleviano momentaneamente il dolore, ma che non rimarginano le ferite e soprattutto non scongiurano le ferite future. Per ultimo l'articolo 3. Il provvedimento disciplina la copertura per opere connesse all'evento della Presidenza italiana del G8. Come al solito, le risorse verranno reperite distraendole dal Fondo per le aree sottoutilizzate, ed in particolare verranno utilizzate quelle già assegnate alla Regione Sardegna a scavalco dei periodi di programmazione. Non siamo così ingenui da indulgere in atteggiamenti ipercritici nei confronti di un evento, la Presidenza italiana del G8, il cui costo potrebbe apparire sproporzionato rispetto alla sua effettiva durata, visto che in fondo si tratta di pochi giorni. Tutt'altro, intendiamo sfidarvi su questo stesso terreno e invitarvi a non lasciare le cose a metà, ma a predisporre ogni sforzo organizzativo ed economico perché questo evento possa costituire davvero una grande opportunità per la Regione Sardegna. Per questo vi preghiamo di prendere in considerazione i nostri emendamenti, che di fatto impegnano e impiegano risorse adeguate alla realizzazione di infrastrutture di collegamento all'evento, nella speranza che possano costituire il lascito più atteso per i territori interessati. Siamo consapevoli che i tempi a disposizione non sono oggettivamente sufficienti alla realizzazione delle opere in questione, ma siamo altrettanto convinti che la situazione di straordinarietà possa costituire una formidabile occasione per definire ambiti di progettazione, affidamento dei lavori e aperture di nuovi cantieri. Un'ultima considerazione proprio sul carattere di straordinarietà dell'evento del G8. Addolora davvero constatare ancora una volta come, in termini di reperimento di risorse adeguate agli impieghi e ai tempi di realizzazione per opere e infrastrutture, questo Paese riesca a rimanere in pari con gli altri Paesi sviluppati solo quando esce dall'ordinarietà delle regole e delle procedure per determinate situazioni di eccezionale straordinarietà. Esemplare a questo proposito è l'esperienza maturata in questi anni dalla Protezione civile, ormai considerata ormai considerata il vero factotum del Paese per ogni evenienza che richieda la normale speditezza realizzativa. Questo è un Paese che ha bisogno di normalità e voi invece tendete ad attribuire a ogni provvedimento il carattere dell'eccezionalità, anche per predisporre interventi o affrontare provvedimenti del tutto ordinari. Vorremmo davvero poter dire di vivere in un Paese normale, dove il Governo si possa far carico dei problemi della collettività

in audizione, non vengono impiegate dove sembrerebbe che invece ve ne sia davvero veramente tanto bisogno.*(Applausi

in seguito all'aumento dei costi delle materie prime energetiche, intende adottare misure di sostegno al settore. Desideriamo esprimere la nostra concordia. Siamo pienamente concordi con il carattere d'urgenza; si tratta infatti di norme che colmano un ritardo un ritardo nell'adempimento previsto dal decreto-legge n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, da attuarsi entro il 30 agosto 2008. Al tempo stesso, voglio anche sottolineare il ritardo nella predisposizione dei decreti di adozione e dei bandi per le procedure di attuazione, previsti, secondo l'articolo 2 del decreto-legge in esame, per il 15 e il 30 novembre del corrente anno. Ciò detto, e premesso che la risoluzione della crisi dei settori dell'agricoltura e della pesca dovuta al rincaro dei costi energetici e petroliferi, nello specifico, deve necessariamente essere inquadrata in un progetto strutturato di interventi e non può certamente esaurirsi all'interno del provvedimento governativo in esame, voglio tuttavia in questa Aula sottolineare che, in sede di discussione in Commissione, con i colleghi del mio Gruppo abbiamo apprezzato e condiviso alcune proposte emendative della maggioranza. Mi riferisco in particolare all'emendamento 2.6, secondo il quale «al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006,

che non venne votato per mancanza del numero legale. Analogamente condivisibili sono l'emendamento 2.300, che prevede, attraverso il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nuovi criteri per rafforzare l'attività dei consorzi di tutela (mi riferisco ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta) e l'emendamento 2.301 in materia di imprenditoria agricola giovanile, che modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, a sua volta ripreso e modificato dall'articolo 1 della legge finanziaria del 2007, commi 1.068 e 1.074. Con tale proposta, al fine di favorire lo sviluppo della nuova imprenditoria in agricoltura attraverso il ricambio generazionale, si prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle agevolazioni di cui al Titolo I, Capo Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. In sostanza, signora Presidente, le tre proposte emendative in definitiva possono essere accolte in quanto riprendono in gran parte il percorso avviato nel corso della XV legislatura ed interrotto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e rappresentano un'opportunità verso la crescita della capacità competitiva del comparto agroalimentare, anch'esso al centro della crisi mondiale finanziaria ed economica che rischia di avere pesanti ripercussioni sui redditi dei produttori, come le stesse organizzazioni professionali sindacali in questi giorni stanno dimostrando. finestra") *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame all'articolo 3 dà attuazione alle previgenti disposizioni legislative relative alla definizione degli adempimenti tributari e contributivi a carico dei soggetti residenti nelle regioni Umbria e Marche che, a seguito della crisi sismica che ha colpito le stesse Regioni nel settembre 1997, hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari

(convertito nella legge n. 103 del 2008) nella parte in cui prevedono che questi soggetti possano definire la propria posizione relativa al periodo interessato alla sospensione corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto di sospensione al netto dei versamenti già eseguiti, in misura ridotta al 40 per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi mediante rateizzazione in 120 rate mensili di pari importo. Il decreto-legge in esame prevede l'inizio della decorrenza delle restituzioni a partire dal gennaio 2009. È evidente che questa misura si pone a coronamento di un percorso legislativo fatto di provvedimenti volti ad agevolare le popolazioni delle zone di Marche ed Umbria colpite dal grave evento sismico del 1997. Soprattutto sottolineo che la riduzione in percentuale delle somme dovute al 40 per cento era volta comunque a garantire che proprio tale restituzione non gravasse in modo insostenibile sui redditi più bassi e sulle imprese. A maggior ragione questa riduzione appare necessaria oggi, che è arrivato il momento della restituzione, visto che gran parte delle medesime zone si trovano a dover affrontare difficoltà economiche legate allo stato di crisi di importanti imprese industriali insediate in quei territori. Da ultimo, vorrei evidenziare un aspetto di fondamentale rilievo, cioè che tale restituzione riguarda, sia per la parte contributiva che per quella relativa ai tributi, tutti i soggetti umbri e marchigiani che a suo tempo beneficiarono delle sospensioni, senza distinzioni tra lavoratori pubblici e privati ed in tal senso, nella prosecuzione dell'esame del decreto-legge, vorrei che si pronunciasse in maniera chiara il Governo anche accogliendo l'emendamento all'articolo 3 da me presentato. A questo punto appare opportuno ricordare, nell'ambito della discussione di questo provvedimento, che a far data dal gennaio 2008 è cessato per le regioni Umbria e Marche lo stato di emergenza proclamato a seguito della crisi sismica. Ciò non significa però che la ricostruzione sia terminata, ma solo che cessa per le due Regioni la possibilità di usufruire degli istituti normativi particolari previsti per gli stati di emergenza. La ricostruzione dei territori si è svolta in tempi brevi, in confronto a casi simili, e rigorosamente entro la stima quantificata subito dopo il sisma. Essa è in avanzato stato di realizzazione: oltre alle abitazioni è stata riparata una consistente parte di opere, infrastrutture ed edifici pubblici e di proprietà ecclesiastica, che hanno consentito la ripresa delle attività socioeconomiche all'interno della vasta area colpita e di ritornare, quindi, alle normali condizioni di vita.

in città e borghi che stanno sorgendo a nuova vita ed impedirebbe la completa messa in sicurezza di alcuni comparti nei centri storici, dove gli edifici sono strutturalmente legati l'uno all'altro; infine, comprometterebbe quel turismo di ritorno che caratterizza i nostri borghi montani, laddove le giovani generazioni, che vivono e lavorano altrove, tornano per passare le vacanze nella casa di famiglia. I finanziamenti ancora occorrenti per portare a termine la ricostruzione sono significativi. Le due Regioni comunque hanno dichiarato nei diversi contesti la disponibilità a ridefinire tale fabbisogno nell'ambito delle risorse occorrenti a chiudere gli interventi di ricostruzione ritenuti indispensabili e, sulla base di questa nuova definizione, costruire una ipotesi pluriennale di chiusura.

mi corre l'obbligo di precisare e di mettere in evidenza alcuni aspetti della vita quotidiana, anche per rappresentare le ragioni della decretazione che mi sembra sia stata oggetto di approfondito dibattito sino a questo momento. Debbo ricordare a me stesso e all'Aula che viviamo un momento di grande difficoltà: una crisi gravissima attanaglia l'Italia, viaggiamo a crescita zero, l'economia è stagnante (è sostanzialmente ferma), i consumi sono ridotti e le imprese sono in grande difficoltà. Ad una situazione di partenza gravissima già al momento dell'insediamento del nuovo Governo nuovo Governo si è aggiunta un'ulteriore crisi finanziaria e bancaria e tutto il sistema è andato in tilt. Questo è, di fatto, il quadro di riferimento in cui si muove ed opera il Governo in un'azione quotidiana di rilancio di attività di sostegno alle famiglie e alle imprese e, in generale, a ciò che occorre per rimuovere dalla stagnazione l'economia nazionale. È vero che si è già affrontata in maniera molto brillante l'emergenza rifiuti e che anche la crisi Alitalia ha avuto un esito positivo. Bisogna richiamare all'attenzione che forse viviamo anche un momento

di impossibilità a gestire i cantieri tanto da portare a richieste di rescissioni di contratti. Se non è emergenza questa e se non si deve intervenire subito con la decretazione, mi domando allora quando si debba intervenire con urgenza. che alcuni emendamenti abbiano portato gli amici dell'opposizione a ritrattare alcune posizioni, accolgo invece con grande positività

alla grande mobilitazione della CGIL, che diventa sempre più sindacato di conservazione, rivolto cioè alla conservazione dei diritti più che allo sviluppo e all'occupazione per proteggere i giovani. A mio avviso, un'opposizione che intraprende una strada dura, sempre più in contrapposizione con la maggioranza, non fa per intero il suo dovere, perché in un momento così grave e difficile serve il contributo di tutti per il superamento dei problemi.

quasi costante e anche a riflessioni comuni, devono poi essere tramite per un'azione di rilancio dello sviluppo, dell'occupazione e dell'economia. Abbiamo bisogno di un momento di grande coinvolgimento: serve maggiore coesione sociale e più impegno da parte di tutti. Credo quindi che, per il senso di responsabilità al quale si fa riferimento nelle more dell'avvento del federalismo, una classe dirigente attrezzata, in grado di assumersi le sue responsabilità,

un confronto sereno che guardi alla soluzione dei problemi della gente, più che a una contrapposizione contro qualcuno. La demonizzazione dell'avversario non ha mai pagato, neanche nelle ultime consultazioni elettorali; occorre, invece, muoversi nella direzione della soluzione dei problemi. penso e spero che anche per quanto riguarda alcuni problemi, tra cui il ritiro dell'emendamento 2.1000, riguardante i fondi FAS, vengano approfonditi seriamente, perché ritengo che una programmazione adeguata possa essere fatta e anche digerita meglio rispetto ad un'imposizione un'imposizione di spesa: parlo di imposizione perché sostanzialmente vengono tolte risorse destinate sicuramente in altre direzioni. *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento al nostro esame rappresenta l'ennesima dimostrazione di come questo Governo non riesca ad individuare gli strumenti necessari per far fronte con efficacia alle urgenze e alle vere necessità del Paese.

ad evitare il blocco delle infrastrutture in Italia, a promuovere lo sviluppo economico nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, a far fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle Regioni Umbria e Marche e, infine, a introdurre disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile.

perché non è pensabile di poter valutare caso per caso tutte le urgenze di questo provvedimento e soprattutto perché, se questo Governo avesse voluto affrontare anche solo un problema di questo Paese (quello delle infrastrutture, ad esempio) non avrebbe previsto nel disegno di legge finanziaria una riduzione delle risorse destinate nel 2009 alle infrastrutture inferiore del 14 per cento rispetto al 2008. Soprattutto, il Governo non avrebbe presentato, e non avrebbe consentito alla propria maggioranza di presentare in Aula e in Commissione, degli emendamenti che nulla hanno a che vedere con questo decreto e che, se approvati in via definitiva da questa Aula, rischiano di stravolgere non solo la natura del provvedimento ma anche l'ordinaria dialettica tra maggioranza e opposizione.

di emendamenti che riguardano l'abolizione *tout court* di tutte le norme introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. che vietano alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti contenenti clausole compromissorie ovvero clausole contenenti ricorso all'arbitrato in caso di disaccordo (mi riferisco all'emendamento 3.0.8 presentato dai senatori Baldini, Zanetta e Grillo); emendamenti che riguardano la reintroduzione dell'istituto della revisione dei prezzi nei contratti dei lavori pubblici; l'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del divieto di arbitrato nei contratti pubblici

e adesso si propone di differirli ulteriormente alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina, applicabile alle controversie arbitrali nei contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture e, quindi, ad una data di riferimento non certa e non individuabile allo stato dei fatti. Insomma, di tutto e di più, per arrivare infine ad un emendamento presentato dal Governo, il 3.0.1, riguardante l'Alitalia e volto a precisare che le disposizioni all'articolo 2112 del codice civile non trovano automatica applicazione, qualora le cessioni di complessi aziendali siano effettuate nell'ambito di una procedura straordinaria di insolvenza. Ebbene, questo articolo del codice civile riguarda il mantenimento dei diritti di lavoratori in caso di trasferimento di azienda. Il vero scopo, lo scopo nascosto di questo decreto sta diventando sempre più chiaro. L'obiettivo che si sta perseguendo è sia quello di continuare a ingerirsi nella questione dei diritti dei lavoratori Alitalia e sia di riportare *in auge* l'applicazione dell'istituto dell'arbitrato nei contratti posti in essere dalla pubblica amministrazione. Di quanto tutto questo costi allo Stato, però, non importa niente a nessuno. La cosa importante è che continuino ad arricchirsi gli arbitri, gli avvocati, tutti soggetti che, non essendo giudici in base alla Costituzione,

Eppure, tutti sanno e lo si è ripetuto più volte in questa Aula che il costo del giudizio arbitrale è sempre stato molto più elevato del giudizio ordinario. Peraltro, le pubbliche amministrazioni, nella stragrande maggioranza dei casi, sono sempre risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri che superano i 320 milioni di euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio, quali i compensi agli arbitri e ai segretari e per il deposito dei lodi. Inoltre, i lodi arbitrali impugnati sono a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della corte d'appello e solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo. Il provvedimento al nostro esame rischia, dunque, di innescare una bomba contro il nostro sistema, per non parlare di tutti gli altri profili rispetto ai quali è possibile sollevare molti dubbi sulla compatibilità costituzionale già evidenziati nella nostra questione pregiudiziale. Intendo sottolineare, infine, che il decreto al nostro esame, oltre a non prevedere alcun finanziamento aggiuntivo a favore delle infrastrutture, dispone pesanti decurtazioni del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), senza chiarire se siano suscettibili di pregiudicare il completamento degli interventi già avviati. Sotto questo profilo, sarebbe utile ricordare al Governo che i fondi destinati al Mezzogiorno non possono sempre compensare il mancato finanziamento ordinario da parte dello Stato dei programmi infrastrutturali. In questo modo, infatti, i fondi FAS perderebbero la loro natura addizionale

Per questi ed altri motivi, che si legano tutti al modo irresponsabile con il quale il Governo sta portando avanti le proprie iniziative, il Gruppo dell'Italia dei Valori preannuncia sin d'ora che esprimerà un voto contrario al provvedimento al nostro esame.

ci vorrebbe un esorcismo, perché, se mai esistesse un genio del male e della cattiva tecnica legislativa, esso si sarebbe annidato e manifestato in questo provvedimento. Ci ha messo del suo il Governo,

un pezzo della giustizia civile, proprio quando stiamo discutendo nelle Commissioni di merito di riforma della giustizia civile), mentre gli elementi che dovrebbero esserci per omogeneità di materia, in questo decreto-legge non ci sono. Ci si è occupati, giustamente, dei terremoti di dieci anni fa, ma si è dimenticato, il Governo, degli interventi urgenti per le alluvioni avvenute in Sardegna meno di un mese fa. Un Governo che guarda all'indietro, ma non è presente nel tempo che dovrebbe utilizzare lo strumento del decreto-legge, che - lo ricordo a tutti - la nostra Costituzione prevede per casi straordinari di necessità e urgenza. [**Presidenza del vice

solo un'inutile litania. Non lo è, colleghi, perché nessuno di noi è esperto di tutto, e chi crede di esserlo non è in realtà esperto di nulla e risulta pericoloso per questo Paese. Ciascuno di noi è assegnato a Commissioni di merito, in cui i problemi possono essere trattati con il concorso delle dovute competenze. Quando queste competenze non ci sono, ci sono gli apprendisti stregoni del diritto (mi dispiace dirlo). È esemplare - non perché sia proposto da apprendisti stregoni, ma perché c'è una pericolosità intrinseca in questo - il caso della reintroduzione degli arbitrati. Sono anni che diciamo che devono finire, che i magistrati devono fare i magistrati e non devono sottrarre il tempo il tempo dedicato alla giustizia pubblica facendo la giustizia privata. Anche il parere della Commissione affari costituzionali, pur se ammantato dalla sapiente prosa del nostro relatore, coperchio per tutte le pentole, il caro collega Lucio Malan, è arrivato a dire di sollecitare la Commissione di merito a valutare l'impatto che l'emendamento potrebbe determinare sul buon funzionamento della giustizia amministrativa, in quanto suscettibile di distogliere una parte dei magistrati dai propri compiti istituzionali. La Commissione di merito ha fatto questa analisi? La Commissione di merito di un problema sulla giustizia e sulla pubblica amministrazione è quella che si occupa dei lavori pubblici o è la Commissione giustizia o la Commissione affari costituzionali? Allora permettetemi di dire, in conclusione, che ci sono delle cose che mancano; una cosa che però c'è, ed è cattiva, è la norma che riguarda il G8 sottoforma di copertura finanziaria di interventi sulla protezione civile. Dopo 34 anni una base militare di sommergibili nucleari va via dalla Sardegna; c'è la possibilità di fare un G8 diverso, testimone di un nuovo tempo della politica internazionale. C'è un accordo tra il Governo e la Regione Sardegna per cui le opere che servono, un terzo, vengono finanziate, è vero, dai fondi FAS, ma quelli interregionali, perché è una questione che riguarda la politica di tutto il Paese. Questo viene scritto dall'onorevole Silvio Berlusconi nell'ordinanza di protezione civile del 31 agosto; il 23 ottobre Berlusconi smentisce se stesso, toglie i fondi Grazie questo G8, che avrà un impatto enorme su tutto il Nord della Sardegna, in un tempo di concentrazione turistica, prevedeva anche la realizzazione di un'importante arteria viaria che improvvisamente sparisce. C'è un certo C'è un certo scimmiottamento da parte della destra della figura del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Credo che dal Mezzogiorno, per questo saccheggio delle risorse già impegnate che gli competevano, dovrà nascere invece una nuova signora Thatcher che, come quella degli anni '80 diceva «*I want my money back*» (io voglio indietro i miei soldi), ricorderà al Governo e a questa maggioranza che le risorse per il Mezzogiorno dovranno essere recuperate altrove. Vi aspettiamo; questa è la sfida!

la realizzazione del piano delle infrastrutture nel nostro Paese rappresenta una sfida concreta, tesa ad avviare un circuito virtuoso fatto di certezze e di prospettive di sviluppo economico, produttivo e occupazionale. Dobbiamo pensare alla realizzazione anche razionale delle opere pubbliche e quando parlo di razionalità intendo che non si può pensare a una grande opera come il ponte sullo Stretto se le infrastrutture che ad esso si innestano sono da Terzo mondo. È come un'autostrada che improvvisamente finisce in un viottolo di campagna; a cosa serve? Mi voglio collegare proprio a questo perché nelle audizioni che abbiamo avuto in Commissione le parti sociali (imprenditori e sindacati) hanno fatto emergere una serie di problematiche sulla difficile situazione di alcuni cantieri (soprattutto al Sud, ma oggi possiamo dire che purtroppo questo sta avvenendo anche in altre parti d'Italia,

e quella dei lavoratori, costretti ad essere sottoposti a ricatti dalla malavita. Riprendiamo l'esempio della Salerno-Reggio Calabria. Dobbiamo tener conto che per realizzare questa infrastruttura ad oggi ha collaborato un'azienda ogni 42 metri. I ritardi intercorrenti dall'aggiudicazione dell'appalto all'avvio dei lavori mediamente superano i 24 mesi in molti appalti, a causa di inadempienze delle vigenti norme di legge, sono stati rescissi gli atti contrattuali. I lavori di alcuni cantieri, a seguito di continui attentati ai mezzi meccanici o alla logistica, subiscono notevoli rallentamenti. A causa delle difficoltà di approvvigionamento di forniture e materiali, nei cantieri in produzione si è in presenza di notevoli incertezze operative. Proponiamo di fare qualcosa che, credo, non riguardi soltanto noi del Partito Democratico e della minoranza, ma anche la maggioranza. Il servizio di alta sorveglianza delle grandi opere dovrà essere territorialmente strutturato garantendo un'unità operativa in ogni prefettura. Proponiamo di consentire al contraente generale il superamento delle percentuali di affidamento dichiarate in sede di gara e agevolarlo affinché lo stesso, laddove produttivamente possibile, reinternalizzi le lavorazioni precedentemente esternalizzate. Per la produzione degli inerti, nei capitolati di appalto, deve essere posto l'obbligo del riciclaggio di materiale proveniente dalle escavazioni. Nei territori dove non è possibile reperire cave che hanno una certificazione antimafia occorre prevedere negli atti di concessione e coltivazione la confisca delle stesse e la nomina di commissari *ad acta*.

così come retribuirli in modo difforme da quello riportato sulle buste paga o, nel caso di avversità atmosferiche, metterli sotto la tutela della cassa integrazione ordinaria e poi obbligarli a lavorare in un altro sito produttivo. i quali la malavita organizzata entra nei cantieri sono prevalentemente quelli del subappalto, della fornitura, della fornitura con posa in opera, dei servizi nei cantieri e dei noli. In molti casi, la malavita organizzata inizia la sua attività ancora prima dell'indizione delle procedure di appalto, oltre a quanto ci è stato detto riguardo la proprietà dei terreni con l'acquisizione delle cave degli inerti, degli impianti di betonaggio. però nella fase della subcontrattazione che la malavita organizzata determina il suo massimo interesse per controllare o tentare di controllare ogni forma di cessione a terzi. Riteniamo che per controllare e governare tutte le fasi del subappaltatore aggiudicatario lo strumento sia quello di applicare la norma del subappalto "di tipo passante" o del pagamento attraverso bonifico bancario. Per quanto riguarda il subappalto di tipo passante, la committente pubblica dovrà indicare nel testo del bando di gara che tutti i pagamenti dovuti dall'appaltatore ai soggetti terzi, erogatori di lavori, di servizio e di forniture, saranno liquidati direttamente alla ragioneria della stazione appaltante. Queste nostre proposte sono importanti se vogliamo far sì che una delle più grandi opere di questo Paese, l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, possa vedere la luce. In questo momento siamo in gravissima difficoltà. Il fatto che possono chiudere cantieri non vuol dire soltanto non realizzare un'infrastruttura, ma non portare avanti una parte del Paese. Ripeto, purtroppo questo sta iniziando ad avvenire in altre parti del Paese. Per scongiurare questo pericolo e raggiungere lo scopo che le opere infrastrutturali si possano e si debbano fare è necessario che lo Stato, in tutte le sue articolazioni, e la società civile lancino una sfida, perché il controllo del territorio non può, non deve e non sarà in mano né agli speculatori né agli individui della malavita organizzata. La Salerno-Reggio Calabria dovrà diventare - se tutti insieme lo vogliamo - un corridoio della legalità. Questa sfida, per essere vinta, deve avere un obiettivo centrale: i lavori devono essere fatti nei tempi, nei luoghi e con i costi convenuti dagli atti contrattuali. Così le infrastrutture diverranno veramente, come tutti vogliamo, volano per rilanciare l'economia del nostro Paese. il Governo con il presente decreto-legge è stato tempestivo nell'affrontare tematiche delicate che interessano il comparto delle infrastrutture, dell'agricoltura, della pesca professionale, dell'autotrasporto e della protezione civile. Tra gli scopi di tale provvedimento, infatti, vi è quello di far fronte alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese e di promuovere Il decreto-legge è strutturato in tre articoli. L'articolo 1 si occupa delle disposizioni in materia di adeguamento di prezzi e modifiche al codice dei contratti, prevedendo per l'anno 2008 l'abbassamento dal 10 all'8 per cento della variazione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi che determinano la compensazione nell'ambito dei contratti di lavori pubblici. Il meccanismo nasce dall'esigenza di intervenire sugli squilibri contrattuali che si sono verificati nel 2008 a causa degli aumenti dei costi di alcuni materiali di costruzione. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l'8 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2008. L'articolo 2 reca norme relative ad interventi di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività di tali settori gravemente compromessi dall'aumento dei prezzi petroliferi. L'articolo 3 è inerente ad interventi in materia di Protezione civile. Le audizioni informali che si sono svolte in 8a Commissione hanno prodotto un'assonanza di vedute e di proposte sul presente decreto-legge da parte dei vari soggetti interessati, sindacati ed imprenditori, come è già stato rilevato anche dal collega Filippi. Dalle suddette audizioni sono emerse numerose questioni. Per ciò che concerne la revisione dei prezzi, il presente provvedimento tratta esclusivamente l'anno 2008 e, quindi, è stata proposta un'azione emendativa volta ad estendere agli anni precedenti le disposizioni introdotte o, per lo meno, a riferire il calcolo revisionale per il 2008 su base trimestrale. Inoltre, le audizioni hanno rilevato che nel calcolo revisionale non esiste il riconoscimento inerente l'incidenza di costo dei prodotti petroliferi e dell'energia che, come è noto, hanno subito notevoli incrementi. La preoccupazione generale emersa è che se il provvedimento non venisse approvato e ulteriormente migliorato le imprese si troverebbero in grande difficoltà in quanto in questi anni hanno subito un incremento di costi delle materie prime di entità molto rilevante, in particolare per ciò che attiene l'acciaio, il bitume e il cemento. Le audizioni hanno altresì evidenziato la difficoltà di alcune imprese, in particolare quelle che operano lungo la tratta Salerno-Reggio Calabria, riferita al problema della infiltrazione malavitosa e tale situazione è stata sottolineata con forza dalle organizzazioni sindacali, le quali hanno manifestato la convinzione che l'infiltrazione malavitosa sia il risultato di una precisa strategia

dovranno essere proposti con urgenza provvedimenti che incidano sulla situazione denunciata che costituisce da sempre una vera e propria emergenza. È stato rilevato come la difficoltà degli enti a corrispondere la revisione prezzi è anche legata al superamento del Patto di stabilità. Altro aspetto sollevato è riferito alle difficoltà connesse con gli *iter* burocratici (conferenza di servizi, procedure di VIA) che rallentano, quindi, l'avvio dei lavori. In considerazione della situazione economica difficile, dove le opere pubbliche diventano un volano importante, si renderà indispensabile intervenire anche in questo settore e ciò potrà essere proposto nel corso dell'*iter* Di grande interesse è stata l'audizione del sottosegretario Bertolaso che ha informato la Commissione relativamente ai lavori di preparazione del G8 presso l'isola della Maddalena, lavori che procedono con un regime speciale e che, a detta del Sottosegretario, risultano svolti in maniera soddisfacente e per i quali questo provvedimento assegna la somma di 233 milioni di euro. Una riflessione opportuna da fare a tale riguardo è che, con procedure accelerate e norme semplificate, anche in Italia si possono realizzare grandi opere in tempi contenuti. Sarebbe quindi opportuno che procedure accelerate possano essere assunte per alcune opere pubbliche condivise dal Parlamento e che sono tuttora bloccate. Il Governo, nella stesura dell'articolo 2 del presente decreto, è andato incontro alle richieste degli autotrasportatori, cogliendo parzialmente le loro esigenze ma, soprattutto, scongiurando la preannunciata manifestazione di protesta. Signor Presidente, in Commissione sono stati presentati una serie di emendamenti che tendono a migliorare il provvedimento. Alcuni di essi sono stati votati positivamente, altri non hanno trovato accoglienza in virtù di difficoltà connesse alla copertura finanziaria. un ringraziamento va al Governo per avere affrontato, con tempestività e incisività, questioni molto importanti su cui vi sono grandi aspettative.

le interrogazioni a risposta immediata in materia di infrastrutture nel Mezzogiorno, con particolare riguardo al ponte sullo Stretto di Messina, previste dal calendario nel pomeriggio di domani, sono rinviate a giovedì 27 novembre, alle ore 15.